il disegno di legge all'ordine del giorno dispone la ratifica di cinque Trattati internazionali, finalizzati alla prevenzione e repressione del terrorismo. Si comprende come il tema sia di estrema attualità e urgenza, considerando la minaccia costante a cui siamo sottoposti già da due decenni. Il terrorismo è considerato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e da ciò consegue che gli Stati parte delle Nazioni Unite devono fare tutto il necessario per contrastarlo. A maggior ragione nel nostro Paese, punto nevralgico degli sbarchi dei flussi migratori nell'area del Mediterraneo, il pericolo del terrorismo risulta essere reale e incombente, per non parlare poi dell'Anno giubilare della Misericordia, un bersaglio troppo ghiotto per tutti quei prepotenti esaltati che utilizzano la religione come strumento di controllo delle masse inermi. Prepotenti esaltati: non c'è altro termine per descrivere chi infanga il nome e la volontà del Padre per giustificare omicidi di massa perpetrati ai danni di ignare vittime da altrettante vittime di un lavaggio di cervello disumano. L'evidenza è infatti fratelli che uccidono altri fratelli in nome di un Dio che niente ha a che vedere con l'unicità e l'unità del Dio degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani, che credono di servire, mentre - in realtà - sono assoggettati, mente e corpo, alla ricerca del potere assoluto dei loro sedicenti capi spirituali. Mi viene subito in mente quanto detto da nostro Signore Gesù contro le cosiddette guide accecate dal potere e dall'esclusività del proprio *status*: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, ottenutolo, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi» (Matteo 23:13-15). Siamo stati testimoni troppo passivi di eventi terrificanti che hanno scosso l'intera Europa e che ci fanno riflettere su quanto l'essere umano sia ancora capace di barbarie dopo secoli di cosiddetto progresso. Non dobbiamo però confondere il giusto impegno nella prevenzione di siffatti crimini contro l'umanità con il rifiuto di ogni e qualsiasi forma di assistenza ai fratelli bisognosi, considerando anche un crimine contro l'umanità e contro Dio qualunque muro o piano di confinamento per liberarci di ospiti sgraditi, perché potenzialmente pericolosi. Mi riferisco, ovviamente, a quanto è successo di recente in Paesi dell'Unione europea molto più civili e democratici del nostro, almeno a quanto dicono. «Allora il Signore disse ad Abramo: "Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per Ma la nazione che essi avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze"». Così si legge nella Genesi biblica (capitolo 15, versetti 13 e 14). La storia del popolo eletto è quella di una stirpe di migranti alla ricerca della casa del Padre, la Terra promessa, ovvero una terra in cui vivere senza colpa,

a fare anamnesi dell'uscita, della fuga, del popolo ebraico dalla violenza degli egiziani. Loro, gli ebrei, i figli di Abramo (nostro e loro padre), ridotti in schiavitù, sfruttati da un popolo che pretendeva di essere superiore, in quanto adoratore di divinità che gli consentivano di dialogare con l'aldilà e di edificare per mezzo delle piramidi la garanzia della sua immortalità. I figli di Abramo, nostri fratelli, considerati un popolo di miseri pastori, adoratori di un Dio minore, andavano sfruttati e maltrattati (secondo la mentalità degli egiziani) ed i loro servigi andavano ricambiati, pagati, con un pezzo di pane duro ed una ciotola d'acqua. Quanti morti, quanta violenza e ciò a causa dell'uomo che sovente pensa di essere superiore, in virtù di credenze teologiche che portano un popolo a considerare il loro Dio migliore,

e distorta, che alcuni esseri umani ed alcuni popoli hanno portato avanti sacrificando milioni di loro fratelli. Colleghi onorevoli, cittadini italiani che ci state ascoltando, ebrei, cristiani e musulmani, voi servitori di un solo Dio, del monoteismo, lo stesso monoteismo del nostro antico e sempre giovane padre Abramo. Lui, Abramo, Abramo, è il fondatore del monoteismo e non lo dobbiamo mai dimenticare. Da Abramo nascerà il popolo ebraico, dal suo discendente Ismaele, figlio di Abramo e della schiava di sua moglie Sara, l'araba Agar, l'Islamismo e da Isacco, frutto della promessa fatta da Elohim ad Abramo e Sara, nascerà il grande Giacobbe e la sua discendenza darà avvio al Cristianesimo. Tre grandi religioni monoteiste; tre grandi fedi, che vanno rispettate; tre grandi popoli, il popolo ebraico, il popolo cristiano e, in ultimo per cronologia storica, il popolo islamico. Tutti e tre figli dell'unico padre terreno: Abramo. Adesso vi chiedo e mi chiedo: possono tutti questi figli dell'unico padre farsi guerra tra loro? Possono massacrarsi? Possono sfruttarsi? Possono non dialogare? Possono non amarsi? Possono non rispettarsi? Basta guerre, basta violenze tra figli dello stesso padre. Non perdiamo di vista ciò che vi ho ribadito poc'anzi, che quasi quattromila nasceva l'Ebraismo e dall'ebraismo, duemila anni fa circa, il Cristianesimo e millequattrocento anni fa circa, l'Islamismo. Tre modi di vedere l'unico Dio, creatore del mondo, del visibile e dell'invisibile, creatore degli universi che ci circondano e di tutti gli esseri viventi che vi abitano, nostri fratelli anche questi ultimi perché creati da chi ha posto in essere tutta l'esistenza. Fratelli e sorelle, figli dell'unico padre e servitore di Dio, Abramo, apriamoci al dialogo e cerchiamo tutti assieme, ebrei, cristiani ed islamici, di trovare un'intesa pacifica che possa dare solo frutti positivi all'umanità tutta Spero che le mie parole, le mie riflessioni e le mie preghiere, possano possano essere motivo e stimolo a livello governativo e diplomatico affinché il tanto auspicato dialogo avvenga. Senza il dialogo non vi può essere futuro, senza il dialogo non vi può essere vita. Pensate al Cristianesimo. Nel Cristianesimo Dio stesso si fa dialogo, Dio stesso sceglie di farsi vero uomo allo scopo di capire come potere meglio dialogare con gli esseri umani. il suo unico figlio, l'Unigenito, sulla terra allo scopo di rinsaldare il dialogo che si era fratturato nell'Antico Testamento, e di preciso nel primo libro del Pentateuco (Genesi),

il dialogo tra Dio e l'uomo viene interrotto, la loro corruzione porterà alla nascita della morte, della malattia, della disperazione, dell'imperfezione, del caos, della mancanza di dialogo tra Dio e l'uomo. Ma dopo quasi due lunghi millenni, Elohim invierà il suo messaggero Gesù Cristo, l'Unto, il consacrato, la sua Parola; il dialogo si farà carne e ciò allo scopo di potere ridialogare con noi esseri umani, allo scopo di ricostruire l'alleanza tra Dio e l'uomo, di redimere i figli di Adamo ed Eva, di mondarli dai loro peccati, di farli rinascere a vita nuova. Il nuovo Adamo, Gesù Cristo, Re e Salvatore dell'umanità, porrà le basi per redimere tutta l'umanità e riammetterla al cospetto di Dio, e condurla così nella Gerusalemme celeste, nel nuovo Eden, nel nuovo paradiso, nell'aldilà. Egli inizia a farci percepire il «già», e nel «non ancora» e nell'escatologia terrena ci prepara continuamente con la Parola di Dio, con il dialogo che, grazie al Verbo fattosi carne, per noi e per la nostra salvezza, ci fa assaporare ciò che poi godremo definitivamente nel cielo. Colleghi onorevoli, amministratori dello Stato, l'umanità ha bisogno di un forte dialogo tra le tre grandi religioni monoteiste e di una legislazione internazionale che possa far capire che tra fratelli l'unica arma da adottare è quella dell'amore. Nel merito del disegno di legge, esso si inserisce nella cornice della cooperazione internazionale in materia di prevenzione e repressione del terrorismo. Il primo dei cinque Trattati oggetto di ratifica è la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. L'Italia l'ha firmata nel giugno del 2005. Il testo della convenzione individua i profili di nuove figure di reato collegate al compimento di atti di terrorismo: si fa riferimento alla pubblica provocazione (istigazione e apologia), alla commissione di un reato terroristico, al reclutamento e all'addestramento ad attività terroristiche che si concretizza nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, nonché di metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici. In tema di provocazione, però, credo di dover aprire una piccola ma doverosa parentesi sul fatto che ritengo profondamente sbagliato anche ridicolizzare la religione, *trend* oggigiorno ampiamente diffuso e spacciato per libertà di parola, arrivando a delle vere e proprie forme di blasfemia inaccettabili, da parte non solo di un credente, ma anche da quegli atei che però professano apertamente il rispetto dell'altrui sensibilità. «Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte: tutta la comunità lo dovrà lapidare. Straniero o nativo del paese, se ha bestemmiato il nome del Signore, sarà messo a morte (Levitico 24:16)». Ovviamente non voglio in alcun modo giustificare la violenza in nome di qualsiasi diritto, compreso quello più sacro della libertà di culto, ma voglio farvi riflettere sul fatto che una semplice ed innocua violenza verbale, in determinati contesti di arretratezza o di povertà, può provocare, anche nelle persone più mansuete, una rabbia che può essere adeguatamente cavalcata e spinta verso direzioni imprevedibili. Dio è speranza e a volte è l'unica ricchezza, quella inestimabile che rimane a chi non ha nulla. E non dobbiamo permetterci di sottovalutare ciò in nome di un cosiddetto progresso culturale che relega la fede a semplice scaramanzia o droga per gli stupidi. «Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo?». Mi riferisco al fatto che l'incitamento all'odio religioso non può essere condannato in un caso e sottovalutato, anzi quasi giustificato, in un altro, perché sempre di odio si tratta e come tale deve essere eradicato su tutti i fronti da quella che vuole considerarsi una società civile. Il secondo è il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, anche se a livello internazionale non è ancora entrato in vigore, perché non tutti gli Stati parte della Convenzione hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati al Protocollo. La terza ratifica riguarda la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Nello specifico, il Trattato amplia la Convenzione del 1990, che disciplina la stessa materia. Adesso, con la nuova Convenzione, sono prese in considerazione anche le forme di finanziamento del terrorismo realizzate attraversa attività lecite. La quarta attiene alla Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York nell'aprile del 2005. Le fattispecie che costituiscono reato connesso ad atti di terrorismo consistono nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni e nel danneggiamento di impianti. Inoltre viene stabilito che anche la sola minaccia di commettere un reato di tal specie costituisce reato, come pure la complicità. Infine si procede alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005. Seppur non ancora entrato in vigore, il Protocollo attribuisce rilievo penale alla partecipazione ad un'associazione a fini terroristici; alla sottoposizione ad un addestramento a fini terroristici; al compimento di viaggi all'estero con finalità terroristiche, al finanziamento di viaggi all'estero di altri soggetti a fini di terrorismo e all'organizzazione e al favoreggiamento in qualunque altro modo di tali viaggi. È previsto altresì il rafforzamento degli scambi rapidi di informazione tra le parti riguardo ai soggetti che si recano all'estero sospetti di essere terroristi. Da un breve *excursus* si evince che tutti gli accordi inseriti in questo disegno di legge per essere recepiti nel nostro ordinamento sono stati firmati quando a Palazzo Chigi c'era il Governo Berlusconi, a riprova del fatto che la conduzione di politica estera del Governo Berlusconi era in piena sintonia con tutti i *partner* occidentali ed era finalizzata alla lotta al terrorismo e alla cooperazione internazionale per contrastare

ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Oggi come ieri il terrorismo colpisce al cuore l'Occidente e i Paesi che si oppongono all'estremismo islamico ed è quanto mai necessario che tutti i Governi convergano verso una strategia chiara e unica per sradicare le cellule e i gruppi terroristici. I Governi sono chiamati a gestire numerose crisi congiuntamente ed è chiaro che l'assenza di una strategia comune alimenta le minacce.

mi sono sentito un po' a disagio, perché non ho capito se eravamo nel Senato della Repubblica o nel Conclave. Quindi, quando mi dirà «*habemus Papam!*» potremo uscire da quest'Aula.

Con riferimento, invece, all'articolo 4 è stata presentata una serie di emendamenti che ha come presupposto una valutazione negativa dell'articolo che ci viene proposto

viene introdotta una nuova figura di reato che prevede la punibilità di una serie di condotte che attualmente risultano già punibili ai sensi della norma relativa al reato di associazione terroristica. Il ragionamento che viene fatto dal proponente è che tali comportamenti necessitino di una punibilità separata in quanto chi li pone in essere non fa parte dell'associazione terroristica pur

Tanto ciò è vero che, dal raffronto tra la norma attuale e quella che si vuole introdurre, le condotte risultano assolutamente identiche, così come identica è la sanzione. Orbene, il reato di concorso esterno si può configurare con riferimento a tutti i reati associativi: si può configurare con riferimento al reato di associazione mafiosa così come con riferimento al reato di associazione terroristica. Nel momento in cui, però, si prevede una disciplina per il cosiddetto concorso esterno in associazione terroristica e non si fa un'analoga operazione con riferimento all'associazione mafiosa, stante il principio di tassatività che governa il sistema penale, noi ci troviamo di fronte alla possibilità, in via interpretativa, che tutto quello che è concorso esterno in associazione mafiosa possa non trovare punibilità per l'assenza di una specifica norma, una specifica norma, la quale invece viene espressamente prevista per il reato di associazione terroristica. E siccome l'interpretazione delle norme si ispira al sistema, con questa innovazione create sostanzialmente un varco non indifferente con riferimento al contrasto mafioso e, in particolare, alla punibilità delle condotte di concorso esterno.

come figure di concorso esterno. È dannosa? Sicuramente sì per gli effetti che essa provoca nel tema del contrasto alla mafia. Liberi voi di decidere come meglio riterrete.

per chiedere - e molto probabilmente per ottenere - la non punibilità di tutti coloro che pongono in essere comportamenti oggettivamente di favore nei confronti dell'associazione mafiosa senza farne parte e che non potranno essere puniti in ragione del principio di tassatività, per l'assenza di una norma specifica che vada a punire quella fattispecie di concorso esterno; norma specifica che invece esiste con riferimento all'associazione terroristica. Dal nostro punto di vista - e sono stati presentati altri emendamenti sul punto - vi sono degli errori tecnici sotto il profilo della quantificazione della pena dell'assoluta parità della sanzione tra la nuova figura e la precedente figura dell'associazione terroristica. Ma se si tratta di una nuova figura, retrogradata rispetto a quella di associazione terroristica, solo perché chi la pone in essere non fa parte dell'associazione terroristica, qual è

di una bomba atomica o di armi chimiche o batteriologiche si possa essere puniti con una pena di quindici

Questa norma è corretta sotto il profilo del sistema giuridico, con riguardo agli atteggiamenti sanzionatori e alla valutazione della gravità dei reati? Sicuramente no.

dall'altra Camera ci pervengono testi erronei. E questo volevamo dirvi, affinché risultasse dal Resoconto stenografico, perché un domani non si venga a dire che la colpa è dei giudici,

di citare cose che in questa sede non sono state dette, o che sono state dette e si afferma essere state interpretate in maniera errata. A voi la responsabilità di indebolire il contrasto alla criminalità mafiosa.

proponendo, introduce una nuova fattispecie di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo al di fuori dell'ipotesi associativa.

ma per un corretto recepimento della Convenzione di Varsavia del 2005, che è il cuore del provvedimento in esame. Quella Convenzione, così come le altre che stiamo andando a recepire, prevede una serie di interventi che, in gran parte, sono già coperti dal nostro sistema penale. In questo caso si tratta di intervenire su alcune piccole misure che, con riferimento a quanto stabilito dalla Convenzione, non sono adeguatamente previste dal nostro ordinamento. In questo caso, per l'appunto, il tema di un finanziamento fuori da una struttura e l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo sono un contesto molto diverso sul piano

dall'articolo 270-*bis* del codice penale, questa è, nel primo caso, relativa a chi partecipa all'associazione e, nel secondo caso, a chi finanzia l'associazione. Quindi, un'equiparazione dal punto di vista della sanzione penale di questi due comportamenti

di diminuire le pene per chi deposita o custodisce denaro: si tratta delle stesse pene che il senatore Cappelletti propone di aumentare.

sia il concetto di beni mobili che immobili che il concetto di denaro. Anche per quanto riguarda l'emendamento 4.7, a prima

di beni o denaro sottoposti a sequestro, chiedo al collega di ritirarlo, altrimenti esprimo parere è contrario. Pure in questo caso, infatti, siamo in presenza di uno degli impegni specifici contratti dal nostro Paese attraverso la stipula della Convenzione di Varsavia del 2005

«Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo», le parole «, al fine di favorirne il proprietario,». Sottolineo il fatto che anche la pena, relativamente lieve, prevista per questa fattispecie di reato, da due a sei anni, non vuole riferirsi alla situazione specifica di chi mette in campo le condotte di sottrazione e sequestro per favorire chi commette la condotta terroristica, azione che sarebbe già punita con pene ben più gravi di questa. Per quanto riguarda gli emendamenti

la sanzione prevista da quella norma per chi crea un ordigno nucleare o ne viene in possesso

Presidente, pur avendo ascoltato con molta attenzione e rispetto le sobrie ragioni di replica del relatore alla proposta del senatore Palma,

delle convenzioni internazionali e, in questo caso, di convenzioni internazionali che hanno come bersaglio il terrorismo. Già, ma le ragioni profonde per le quali tocca all'Aula del Parlamento ratificare i trattati internazionali sono quelle di poter constatare che i reati contro la personalità dello Stato sono estranei alla cultura democratica, alla cultura dello Stato liberale e dello Stato di diritto. Per quanto riguarda più specificamente la guerra contro il terrorismo, vorrei ricordare a quest'Aula che il nostro Paese, il nostro ordinamento giuridico, pagando un prezzo altissimo, hanno lottato con la propria magistratura, con le proprie Forze dell'ordine, con i propri esponenti politici contro il terrorismo, senza mai calpestare gli ideali dello Stato di diritto. Per cui l'improprio richiamo allo Stato etico, se non vogliamo dire alla continuità dell'ordinamento fascista in sede di ratifica dei trattati internazionali, è un modo di calpestare le ragioni, le vite umane e i costi di lealtà all'ordinamento costituzionale che allora pagammo. Di qui la necessità di approvare - a mio giudizio - l'emendamento proposto dal collega Palma.

una problematica che può essere giusta o sbagliata, ma qualcuno mi dovrebbe spiegare perché è sbagliata. Si costruisce un sistema squilibrato per cui si tipizza nel codice penale

può capitare che l'armamentario antimafia e anticriminalità organizzata costruito decada nel momento in cui norme specifiche disciplinano - come in questo caso avverrebbe - il concorso esterno in questioni che riguardano il terrorismo. Qualcuno ha risposto?

Mi domando se il Senato possa discutere di questioni di una tale importanza e spessore senza che nessuno sia in grado di difendere una posizione che viene proposta

Allo stesso tempo si aprono scenari interpretativi e applicativi delle norme giuridiche che, in futuro, ci potrebbero portare a riconoscere che in questo momento stiamo commettendo un errore. Qualsiasi distorsione o equivoco che possiamo introdurre

si legge: «Chiunque sottrae... beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo». Le condotte con finalità di terrorismo hanno giustificato il sequestro. Non è la finalità del ladro che sottrae i beni e il denaro.

La volontà dell'opposizione è di migliorare il testo e rendere più efficace la lotta al terrorismo sotto il profilo di norme che hanno un loro significato specifico e che non possono essere dubbie. Nella

allora individuammo - lei lo ricorderà, Presidente - al Consiglio superiore della magistratura, su proposta di Michele Coiro e del sottoscritto, una sola aggravante

che ci troviamo di fronte a un atto già approvato dalla Camera. Si può cambiare un atto approvato dalla Camera? CALIENDO *(FI-PdL lo abbiamo fatto tante volte. Non vi è, quindi, nulla di scandaloso nella proposta che viene avanzata di approvare emendamenti che modificano un atto già approvato dalla Camera. Noi ci appelliamo alla necessità di approvare un atto del Senato che sia conforme a quello della Camera, a prescindere da una valutazione di merito

ma anche coerenti con le convenzioni internazionali che abbiamo il dovere - direi l'obbligo - di recepire nel nostro ordinamento, come chiede la nostra Costituzione. Presidente,

grazie al lavoro svolto in tanti e tanti anni all'interno del nostro Paese, ma debbo dire anche grazie alla capacità del Governo di essere in allerta, pronto, vigile

Queste forme di condotta sono novità che l'apparato codicistico, spesso dell'Ottocento, non è in grado di prevedere. Cari colleghi, le nuove condotte da terrorismo

la confisca dellecose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto». Questa è un'altra importante condotta da colpire,

la personalità interna dello Stato la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare. La disposizione di cui al comma 1, lettera *c)*, punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque, con finalità di terrorismo, procura a sé o ad altri materia radio-attiva, crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Questi sono i contenuti dell'articolo 4. 4. Con riferimento alle prime due condotte (ossia colpire chi raccoglie o mette a disposizione denaro con finalità di terrorismo, al di fuori della sua appartenenza all'associazione terroristica, che è la caratteristica del terrorismo globalizzato),

del senatore Palma è quella di preservare sul piano giurisprudenziale la possibilità di colpire il concorso esterno.

sono le stesse previste nel 270-*quinquies*: associazione terroristica. La differenza tra le due norme, quella vecchia e quella che si vuole introdurre, è che il soggetto che pone in essere le condotte di cui alla norma che si vuole introdurre non fa parte dell'associazione terroristica. Alla luce di una giurisprudenza consolidata in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, si sta disciplinando il concorso esterno in associazione terroristica. Lei, signor Presidente (come me e come tanti altri), sa perfettamente che il concorso esterno in un reato associativo può essere configurato con riferimento all'associazione mafiosa, ma anche con riferimento a tutti gli altri reati associativi. Le condotte, quindi, che si vogliono introdurre con una nuova punibilità - peraltro con la stessa identica sanzione dell'associazione terroristica - sono le stesse della associazione terroristica.

l'eventuale reato di concorso esterno in associazione mafiosa potrà essere aggredito sul piano interpretativo-sistematico, perché nel campo dell'associazione mafiosa manca una specifica figura delittuosa che invece è prevista per l'associazione terroristica. È questo il punto che volevo mettere in evidenza. chiedendo: questa norma è utile? Non lo è, perché dette condotte sono già punite con la stessa identica sanzione secondo la norma attuale.

Ho ascoltato la replica del relatore e non voglio fare polemica, ma una me la consentirà il senatore Lumia, che probabilmente è stato disattento: il nostro codice penale, a dire la verità, nel suo

gli emendamenti sostanzialmente dicono che noi non siamo d'accordo per le ragioni che abbiamo espresso. Volete introdurre questo reato? Benissimo, ma non potete prevedere la stessa pena dell'associazione terroristica, terroristica, altrimenti violate il principio di ragionevolezza. Avete immaginato delle altre figure per un impossessamento di beni sequestrati al fine di favorire il proprietario, ripetendo peraltro la norma già presente nel codice?

Siccome nel nostro sistema penale vige il principio della tassatività, come avete fatto per il 270-*sexies*.1, non era forse il caso di aggiungere «salvo che non ricorra il reato di cui agli articoli 200 o 270 (e via dicendo), la pena è questa»? Come vede, al fine di favorire il proprietario,

Pepe)*. Signor Presidente, per essere chiari, questo è il senso dell'intervento che mi sono permesso di fare - ripeto - stante la sua presenza in Aula, della quale - ripeto - sono contento. Noi non abbiamo presentato emendamenti ostruzionistici all'articolo 4. Abbiamo immaginato di contribuire al lavoro del legislatore ponendo una serie di problemi che non possono essere superati in politichese. Ci dovete rispondere sul piano tecnico, e fino ad ora risposte sul piano tecnico non ce ne sono state. Signor Presidente, conviene con me - non dico che sia certo, ma che sia possibile, forse estremamente probabile - che possa avvenire sul piano interpretativo quello che dico io? Conviene con me che il sistema sanzionatorio dei reati per terrorismo non può essere sganciato dal sistema sanzionatorio Volete andare avanti con questo provvedimento? Andate avanti. Non volete scontentare la Camera e i *mantra* della Camera? Non fatelo. Però consentite - non si può fare una discussione sul terrorismo e sulla criminalità mafiosa parlando singolarmente per Gruppi ognuno dei fatti propri e senza dare ascolto a nessuno. Signor Presidente, le sarei grato se volesse consigliare l'accantonamento dell'articolo 4 e di tutti gli emendamenti relativi a tale articolo, per consentire non dico sul piano tecnico - ormai non ho più alcuna fiducia in questo - ma almeno sul piano politico, un ragionamento alla maggioranza.

da parte di chi non fa parte dell'associazione terroristica è già punito con la stessa pena che voi indicate ai sensi della norma attuale. attuale. Non c'è bisogno di queste operazioni, che creano solo confusione e costituiscono meri e - mi consenta - abbastanza squallidi *spot* pubblicitari. Chiedo pertanto che venga accantonato l'articolo 4 e tutti gli emendamenti

la preoccupazione del collega è quella di vedere tipizzato il reato di concorso esterno in associazione terroristica, laddove nel nostro sistema non vi è una figura già tipizzata del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. mafiosa. Per la verità, essendo da sempre un sostenitore della certezza del diritto, anche sotto il profilo della qualificazione delle condotte delittuose, avrei auspicato che nel nostro Paese ci fosse stata una norma che tipizzasse, appunto, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in considerazione del fatto che esso è di derivazione giurisprudenziale e si presta talvolta

un'attività delittuosa vi è la previsione tipizzata del concorso esterno, ben può essere di conforto a quell'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel nostro Paese.

della ragionevolezza e dell'equilibrio delle sanzioni per le singole figure delittuose, non ci può non essere un'equilibrata commisurazione. Per cui non è immaginabile - il senatore Lumia non c'è più, se n'è andato, ma è presente Lo Giudice - che vi sia una previsione di pena identica sia per il reato di terrorismo che per il reato di concorso esterno. Questo sì contrasta con l'attuale giurisprudenza italiana in tema di concorso esterno in associazione camorristica, tant'è che le pene lì sono differenziate.

signor Presidente, al fine di consentire una maggiore riflessione non già sulla prima questione, ma piuttosto sulla quantificazione delle pene per le varie figure che si vanno ad introdurre, invito invito il relatore e il Governo ad una riflessione su questo punto ed eventualmente mi associo alla richiesta di accantonamento. Diversamente, gli

ho ascoltato anch'io con attenzione quanto esposto dal senatore Palma e dagli altri colleghi che sostengono l'opportunità quanto meno di accantonare l'articolo 4, con riferimento ai rilievi sollevati dal senatore Palma, relativi all'inutilità e addirittura alla dannosità che la norma potrebbe introdurre nel nostro ordinamento, per quanto riguarda la questione dell'articolo 416-*bis* e l'attuale situazione giurisprudenziale sulla contestazione del concorso esterno.

che prevede il reato di associazione. Quindi, con la specifica normativa già esistente, si tratta di condotte che si pongono al di fuori dell'ambito associativo e quindi anche del concorso. A me sembra che la punizione del mero finanziamento, ad esempio nei confronti di chi svolge attività di addestramento o di arruolamento, con la specifica che il finanziamento riguarda le condotte con finalità di terrorismo, non possa creare dei pericoli interpretativi o addirittura di estensione analogica *in bonam partem* per chi

rispetto alle varie ipotesi di reato già previste nel nostro ordinamento, che si pongono al di fuori delle ipotesi associative, ma anche di concorso.

successivi sul terrorismo nucleare. Porre la disposizione per cui la reclusione non debba essere inferiore a 15 anni, a fronte della possibilità di punire in maniera molto più severa, con un tipo di pena diversa qual è l'ergastolo, chi utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare mi pare francamente un'osservazione giusta, tanto più se teniamo a mente quanto abbiamo votato l'anno scorso in tema di diritti ambientali, quando, seppur con pene molto severe, abbiamo punito con un massimo forse di quindici anni chi si rendeva responsabile di disastro ambientale.

osservazioni su due delle questioni emerse nelle dichiarazioni di voto. La prima riguarda di nuovo il tema dell'intromissione della norma che noi andremo ad approvare con

ma spesso presenta forme del tutto nuove e inafferrabili con azioni che, commesse con finalità di terrorismo, mostrano deboli legami con una struttura associativa. È di questo che stiamo parlando, ed è quindi su questo che c'è la necessità d'intervenire per poter colpire chi attui di fatto un comportamento a terrorismo, ma non attraverso una individuabile e comprovabile appartenenza strutturata a un'associazione. Per quanto riguarda la questione inerente agli ordigni nucleari,

nelle dimensioni plasticamente prima rappresentate, ma di una gamma di comportamenti che possono arrivare laddove si innestano anche altre fattispecie di reato, nel caso in cui si utilizzi una bomba nucleare. Ciò riguarda anche quei comportamenti che possono essere

Pertanto, rispetto alla richiesta di accantonamento, signor Presidente, io propongo di proseguire con le votazioni sull'articolo 4 e sui relativi emendamenti.

prima delle parole «mette a disposizione beni», le parole «deposita, custodisce, intermedia»

cinque a dieci anni verrebbero sanzionate con la pena prevista dal comma precedente. Questo è il motivo per cui quella che poteva sembrare o poteva essere nelle intenzioni dei proponenti una semplice specificazione, in realtà, ha l'effetto di un aumento di pena.

molte associazioni o gruppi di persone raccolgono fondi da destinare a persone danneggiate dalla guerra nei teatri mediorientali. Con queste somme danno aiuto a popolazioni che sono assolutamente abbandonate dalla comunità internazionale. allora non formulare in termini meno che chiarissimi questa norma, così come mi pare sia fatto,

recanti tale specificazione, rappresentano un timore in sé condivisibile, ma che non ritengo possa essere considerato effettivamente riconducibile ad un rischio derivante dalla formulazione in esame. È evidente che stiamo parlando del finanziamento di condotte con finalità di terrorismo diamo per scontato il fatto che ci sia una intenzionalità e una conoscenza inequivocabile della finalità per cui quei soldi verranno utilizzati.

Ho trovato la piena conferma (che era superflua, probabilmente, perché sono termini che tutti noi conosciamo e utilizziamo quotidianamente) rispetto al fatto che la parola «fondi» contenga in sé

quindi, l'utilizzo della parola «fondi» all'interno dello stesso articolo che utilizza, in altre parti, le parole «beni o denaro» deve essere inteso come l'utilizzo di un termine sicuramente e completamente sinonimo

la legge che voi state per votare dice che chiunque, come atto di terrorismo, faccia parte di un'associazione terroristica, crei e quindi detenga un ordigno nucleare, è punito con la pena da sei a dodici anni.

nucleare? La detenzione di un'arma da guerra particolarmente micidiale ha una pena leggermente inferiore rispetto a questo. questo. Siccome il sistema sanzionatorio si ispira a criteri di ragionevolezza, voi ritenete ragionevole che il terrorista che ha un ordigno nucleare e che, evidentemente, lo possiede non come soprammobile ma perché nella sua testa evidentemente ne immagina un futuro utilizzo, debba essere punito con una pena da sei a dodici anni? Così come successivamente così facciamo contento il senatore Lo Giudice - lo stesso terrorista, che quell'ordigno nucleare utilizza, viene punito con una pena non inferiore ad anni quindici. Benissimo, siamo d'accordo. Ma se un terrorista detiene un ordigno nucleare, invece della pena da sei a dodici anni immaginiamo una pena non inferiore ad anni

possono nascere effetti meno devastanti di un omicidio? E se, parlando di ordigni nucleari, la cosa vi sembra impossibile, immaginate allora tutte le armi chimiche e batteriologiche che possono essere tranquillamente, per fini terroristici, detenute e utilizzate. Pertanto, voi ritenete che vadano bene queste pene? Votatele; però ricordo a tutti voi che la pena ha anche un effetto di deterrenza, e se il possesso di un ordigno nucleare prevede nel minimo la pena di sei anni, in ragione dei vari meccanismi di alleviamento della pena che ci sono all'interno del nostro codice, non venite poi a lamentarvi e vi invito a non fare polemiche nei confronti dei giudici se per ipotesi, a fronte del possesso di un ordigno nucleare, vi troverete di fronte a una pena magari di anni quattro e

del senatore Palma, mi pare strano che qualcuno possa non condividere dei ragionamenti così semplici ed elementari. PRESIDENTE. Senatore Palma, autorizza il collega alla sottoscrizione dell'emendamento? Con grande piacere, anche perché lo utilizzo come ringraziamento per il modesto contributo fornitomi prima. in dissenso dalla posizione del mio Gruppo e non intendo partecipare al voto perché reputo ridicolo che il relatore e i membri della Commissione non si fermino di fronte a questo scempio del diritto che si sta facendo. Stiamo ridicolizzando il Senato e offrendo argomenti per la sua abolizione, perché trattare meno degli incidenti stradali l'uso di ordigno nucleare è veramente incredibile. Signor Presidente, faccio appello a lei poiché, essendo stato Presidente della procura antimafia, che adesso è diventata

che negli ultimi anni è soprattutto guidato da motivazioni religiose, nella gran parte dei casi è un terrorista *kamikaze*, un terrorista suicida. Questo tipo di riflessioni, come quelle del presidente Palma, hanno una consistenza in un pensiero, in un modo di ragionare occidentale, quello per noi usuale. Nel caso di terroristi disposti a generare una deflagrazione nucleare

ma essa deve anche saper configurare uno scenario. Sul piano prettamente politico, immaginare che ci sia una pena che convince e attira chi è nelle condizioni di detenere un'arma nucleare è realmente irragionevole.

a riflettere su quello che stiamo facendo. È come se stessimo dicendo: investite in armi nucleari in Italia e detenetele in Italia perché, facendolo, vi

reato. Nessuno è così matto da pensare che chi produce una strage attraverso l'utilizzo di un ordigno nucleare potrà essere punito con un massimo di ventiquattro anni. È evidente che non è così. non è così. Stiamo ragionando di uno scenario diverso da quello effettivamente prodotto da questa norma, che interviene, invece, su dei comportamenti specifici punendoli in modo specifico per quello che sono. Mi riferisco alla cessione, alla detenzione e al danneggiamento di un ordigno nucleare che crei il rischio di emissione di materiale radioattivo.

ciò che emerge e sgomenta è il dato politico: il rifiuto di questa maggioranza di ascoltare qualsiasi consiglio

non voler dialogare su nulla. Penso una cosa e quella è. O prendi questo o te ne vai a casa. Ci rendiamo conto? Sembra un'esagerazione, ma questi comportamenti portano a dire: ma che stiamo a fare qua? senatore Pepe)*. Veramente vorrei dire quella maledetta parola: Aventino. Non serve a niente parlare con serenità, dialogare e confrontarsi. No, questo è

un po' di coraggio da parte di tutti, un po' di presa di coscienza del proprio io, delle proprie idee e della propria dignità.

Presidente, il diritto penale, anche con riflessi internazionali, non può essere nelle mani di relatori così incompetenti. Propongo l'accantonamento di questo provvedimento, perché con il diritto e la lotta al terrorismo non si scherza e non si gioca. Sospendiamo l'esame di questo provvedimento.

è evidente che alla luce dell'approvazione dell'emendamento

Presidente, credo sia ragionevole accedere alla richiesta avanzata dal senatore Palma,

Il senatore Lo Giudice ha illustrato con completezza, esattezza

imballata sulla discussione di un emendamento, una volta ottenuto il risultato, si è alzato e ha detto: «Avete visto? Adesso dobbiamo ridiscutere il provvedimento, adesso il provvedimento non ha più senso».

le chiedo, per cortesia, di accedere alla richiesta del senatore Palma e, per un tempo ragionevolmente breve, di concedere la sospensione immediata dei lavori dell'Assemblea*. Signor Presidente, vorrei ringraziare il presidente Zanda per avere acceduto alla mia richiesta, anche se oggettivamente non riesco a comprendere a quale richiesta egli abbia acceduto, se a quella vera (fermiamoci quindici minuti per ragionare su questi due emendamenti e capire quale dei due deve avere il parere favorevole del relatore, ovvero su un eventuale ulteriore emendamento del relatore in materia) a quella, sicuramente non vera e che rientra nella fantasia del senatore Zanda, ossia che io avrei chiesto di ridiscutere integralmente l'intero provvedimento. Un'ultima cosa, signor Presidente. Credo che in quest'Assemblea, nei limiti consentiti dalla politica e dalle anomalie della politica, abbiamo il dovere di dire fino in fondo la verità.

Abbiamo sollevato anche in quest'Assemblea una difficoltà nella quale ci troviamo da tempo, da parecchi mesi, generata dalla impossibilità di avere gli spazi e i tempi per poter discutere in modo adeguatamente approfondito dei provvedimenti che sicuramente sono complessi. È vero anche quanto afferma il senatore Palma: la Commissione giustizia, esattamente come il Senato, è una Commissione nella quale il peso della maggioranza è determinante per l'andamento dei lavori stessi. Ci siamo visti sottrarre anche provvedimenti che sarebbero stati di competenza della Commissione giustizia, riunita con altre; abbiamo sollevato un conflitto di attribuzione e abbiamo cercato di evitare

che appartiene esclusivamente alla maggioranza sembra veramente ingiusto nei confronti di chi comunque intende lavorare seriamente. Signor Presidente, non vorrei essere pedante, ma ci tengo a dire che quanto è accaduto stamattina è un caso di studio da portare all'attenzione

e apporta ulteriori significati e ulteriori argomentazioni rispetto a quanto avvenuto in Commissione. mi pare sia avvenuto questo. L'intervento del collega Tarquinio è stato in qualche modo un appello all'Assemblea a riprendersi le sue competenze. In questa legislatura abbiamo visto Commissioni sbarrate che non hanno discusso i provvedimenti; abbiamo assistito

dovere dobbiamo anche sentirci dire che è una deviazione o una prepotenza. Un Parlamento funziona esattamente come abbiamo visto stamattina, e su questo credo che le lezioni possono esserci risparmiate e soprattutto possono essere risparmiate al Paese. Finalmente oggi abbiamo dato un esempio di dignità. *(Applausi

Non concordo con Zanda rispetto al ruolo delle Commissioni: le Commissioni hanno un ruolo preparatorio, ma il passaggio in Assemblea è quello definitivo e finale.

Domenica ci sono stati i ballottaggi, che sono andati in una certa maniera. Domani c'è la direzione del Partito Questa è la prima volta che il Governo, con un voto palese, va sotto, perché tutte le volte si erano modificati i pareri rimettendosi all'Assemblea. Oggi per la prima volta, con il voto palese, maggioranza e Governo vanno sotto. Quindi, ovviamente, si è visto quest'oggi quello che accadrà in futuro: quando la barca affonda, i topi scappano. I voti contrari all'emendamento sono stati quelli ortodossi, cioè i voti del PD; i voti delle "ali" e delle "alette" si stanno squagliando, perché la nave affonda. Tanti auguri; stia sereno il Governo Renzi e così la sua maggioranza.

pensavo di essere stato estremamente chiaro nel mio intervento quando ho chiesto un momento di riflessione: di un momento di riflessione affinché il relatore potesse, se del caso, cambiare il suo parere in ordine ai due emendamenti, ovvero presentarne uno nuovo.

si assuma la responsabilità, in una materia così delicata, di esprimere il proprio pensiero attraverso un parere: parere favorevole a questo emendamento; parere contrario a quest'altro emendamento. E poi l'Assemblea voti come voti. Quindi, evidentemente, signor Presidente, non ho alcuna intenzione di ritirare i due emendamenti per lo stesso ragionamento fatto dal senatore Caliendo. Da vecchio frequentatore (ahimè, troppo vecchio) di queste Aule parlamentari, se mi è consentito, io alla maggioranza vorrei dare un consiglio: non deve fare gli accordi con noi ma con il Gruppo di AL-A, se è vero come è vero che fino a quando il Gruppo di AL-A ha votato con il Governo gli emendamenti sono stati respinti e appena il Gruppo di AL-A ha votato in modo dissonante dal Governo e dalla maggioranza l'emendamento è stato approvato. Il che, evidentemente, diciamocelo francamente, pone un problema politico serissimo:

allora il momento di uscire dall'equivoco. O li fate entrare al Governo (apro e chiudo una parentesi: segnalo per un incarico governativo il mio amico, senatore Falanga) ovvero la finite con l'ipocrisia ed evitate di dire che i voti di AL-A si aggiungono. I voti di AL-A sono per voi determinanti!

precisare che io sono un sostenitore leale del Governo e di questa maggioranza, ma mantengo, come riferimento principale, la mia autonomia di giudizio rispetto al merito delle norme proposte in quest'Assemblea. Credo che questo ragionamento lo abbiano fatto altri colleghi della maggioranza, del mio Gruppo e anche di altri Gruppi, non escluso il Gruppo di maggioranza relativa, che hanno ritenuto sul punto di condividere l'emendamento

al primo firmatario dei due emendamenti e accordandoci dopo sul fatto che avremmo potuto convergere sull'emendamento 4.12, attraverso il previo ritiro dell'emendamento 4.13,

richiedere pene elevatissime, stabilire la pena fissa dell'ergastolo per chiunque, in maniera generale e generica, utilizzi un ordigno nucleare con il pericolo che rilasci

e della configurazione di reati di una pesantezza assoluta, non si possa determinare un ambito di discussione che trascende il merito e sconfina nelle vicende politiche e di tenuta della maggioranza al

consolidato di questo Parlamento che affronta questo tipo di questioni prevalentemente attraverso l'aumento delle pene, in una situazione che riguarda questo Paese che vede una certa condizione del sistema carcerario e del sistema della giustizia, privati dei privati dei mezzi necessari per assolvere pienamente al proprio compito. Penso che fare un'operazione politica su questi argomenti non sia una cosa giusta e neppure sopportabile. Noi ci asterremo su tutti i due gli emendamenti, perché ci vogliamo astenere da questo modo di affrontare i problemi. Io non ho apprezzato, seppure le argomentazioni che sono state rappresentate hanno un'assoluta dignità, il fatto che si sia utilizzato questo strumento

che riguardano la vivibilità dei rapporti di maggioranza interni fra forze politiche. Per questa ragione, e solo per questa, noi ci asterremo dal voto di questi due emendamenti.

Sono rimasto soddisfatto delle spiegazioni date dal relatore Lo Giudice rispetto all'emendamento 4.12, quindi l'invito che faccio ai colleghi Palma e Caliendo è di procedere al ritiro dell'emendamento 4.13

In Commissione siamo disponibili come forza d'opposizione tecnica a dare sempre un ausilio e un contributo.

non sia sufficiente. Penso che sia condivisibile sostenere la tesi originaria dell'emendamento 4.13, che a questo punto faccio mio. Al di là degli infingimenti e delle tattiche politiche, dopo aver preso atto che i voti del del Gruppo di AL-A e anche di molti senatori della maggioranza del Nuovo Centrodestra sono stati sfavorevoli al Governo e lasciando *a latere* ogni considerazione di tipo politico sulla maggioranza che sostiene questo Governo in occasione dell'emendamento che è stato votato poco fa,

dialettica tra le parti, votare contro il parere del Governo e del relatore fosse nelle possibilità e nelle giuste dinamiche di svolgimento dei lavori dell'Assemblea. Il fatto che si sia creato un

difforme lo trovo gravissimo. È un segno molto grave di un decadimento degli istituti democratici.

incriminato di fatti di reato, rispetto alla figura più attenuata dell'agente sotto copertura, cioè dell'infiltrato, l'agente che non provoca il reato, ma si inserisce negli ambiti associativi o nelle configurazioni criminose al fine di facilitare l'emersione dei fatti di reato.

ci tengo che rimanga agli atti che quest'Assemblea voterà a favore di una figura che, in astratto, è stata molto contrastata quando si parlava di corruzione.

che una figura in un contesto ha un ruolo e produce delle conseguenze, mentre in un altro contesto e per altri fini ha tutt'altro risvolto, per cui di fatto non sono figure sovrapponibili. Pensiamo alle conseguenze e all'interpretazione che può essere data a una figura strumentale

Apprezzate le circostanze,

ricorrerà il trentaseiesimo anniversario del disastro aereo di Ustica senza che si sia raggiunta una verità univoca e condivisa sull'accaduto. Abbiamo recentemente scoperto che importantissimi documenti classificati come segreti e segretissimi, che abbiamo potuto consultare come membri della Commissione di inchiesta sull'assassinio di Aldo Moro ma la cui divulgazione dopo trentasei anni è ancora penalmente perseguibile - contengono preziose indicazioni per spiegare le cause dell'esplosione dell'aviogetto. Abbiamo sollecitato il Governo a desecretare questi atti, perché l'opinione pubblica e i familiari delle vittime hanno il diritto di conoscere le minacce di rappresaglia su vittime innocenti avanzate ripetutamente dal fronte popolare per la liberazione della Palestina manovrato dai libici nel maggio-giugno 1980, sino ad identificare un aereo possibile obiettivo della rappresaglia stessa. La pubblicazione di questi atti può dare un contributo decisivo per sfatare anche ipotesi da fantascienza e depistaggi che hanno avvelenato la storia di questo disastro aereo.

giugno il Capo dello Stato, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera faranno un appello a conseguire la verità, al di là di ogni convenienza. Quindi, perché questa si persegua, bisogna che il Governo, dopo trentasei anni, pubbliche queste carte e lasci agli storici, all'opinione pubblica, ai magistrati, la possibilità di farsi un'opinione su una situazione ancora oggi aperta, che ci vede in conflitto con gli Stati Uniti, con la Francia, e che inevitabilmente dovrà avere una condivisa e univoca

Tutti sicuramente ricordano le immagini dei paesi straziati: Mirandola, Medolla, Cavezzo, Finale Emilia, San Felice sul Panaro e molti altri borghi. Fu un disastro per vite perse e distruzione. Per gestire l'emergenza e provvedere alle varie fasi legate alla ricostruzione, la pubblica amministrazione si è avvalsa anche di lavoratori somministrati. La Regione Emilia-Romagna, insieme con l'agenzia Obiettivo lavoro, prima, e Manpower, adesso, non ha programmato un percorso formativo *in itinere* per ciascun lavoratore in modo da facilitarne la ricollocazione lavorativa, una volta conclusa l'emergenza terremoto. Eppure, sono state messe a disposizione competenze di ogni tipo, con esperienze professionali di rilievo. Con l'uso smodato dei lavoratori somministrati, la pubblica amministrazione dimostra di concorrere alla precarizzazione del lavoro, dando l'idea che possano esistere dei lavoratori usa e getta. La formula è sempre la stessa: «Ti prendo, ti sfrutto finché mi servi, ti faccio svolgere un lavoro pari a quello degli altri dipendenti, ma non ti riconosco le garanzie sul lavoro, e soprattutto, una volta che non ho più bisogno di te, ti mando a casa». È chiaro che se un lavoratore si trova in questa situazione sarà sempre ricattabile, ostaggio dell'arbitrio del dirigente piazzato dal politico di turno. I lavoratori interinali diventano così merce di scambio politico e ciò vale sia per i lavoratori di "Sisma Emilia" che per tutti gli altri. Non risulta etico utilizzare un impiegato, con le modalità che sono state assegnate nell'ambito della ricostruzione, più di quindici-diciotto mesi senza offrire in cambio una una qualche prospettiva di impiego o almeno di riutilizzo delle competenze maturate. Ad oggi, le funzioni svolte dai somministrati all'interno degli enti locali rappresentano l'ossatura l'ossatura portante di molti uffici (ricevimento del pubblico, interfaccia con i professionisti esterni, sopralluoghi nei cantieri); attività che prima del sisma del 2012 non erano previste neppure per il personale di ruolo. Pertanto, è probabile che molte assunzioni abbiano avuto il solo scopo di utilizzare il personale per far fronte alle mancanze di organico per le attività ordinarie o per smaltire il lavoro arretrato. Data la delicatezza del tema, ho inoltre depositato un atto di sindacato ispettivo

Signor Presidente, era il luglio 2013 quando ho cominciato a raccontare le vicende della comunità Il Forteto.

Noi abbiamo presentato un disegno di legge per istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare, perché vogliamo andare a fondo. È la stessa conclusione cui sono arrivati i membri della commissione d'inchiesta della Regione Toscana: commissariamento della cooperativa cooperativa Il Forteto, perché ancora coinvolta con le vittime e con i carnefici di questi fatti assurdi ed atroci. Invito quindi tutti i parlamentari toscani a a farsi carico di questa Commissione d'inchiesta parlamentare e a sottoscrivere il testo depositato a mia prima firma, l'Atto Senato 2093, per mettere finalmente la parola fine a questa tragedia, che ha colpito non solo le vittime, ma tutti i cittadini toscani e italiani, perché è una vera vergogna quella